L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunico che in data 21 settembre 2017 il Presidente del Senato e la Presidente della Camera dei deputati hanno proceduto alla nomina dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, di cui alla legge 17 luglio 2017, n. 107. L'elenco dei componenti sarà pubblicato in Allegato al Resoconto della seduta odierna. La Commissione è convocata per la sua costituzione domani, mercoledì 27 settembre 2017, alle ore 14,30, presso l'Aula del quarto piano di Palazzo San Macuto, in via del seminario.

dopo l'illustrazione delle mozioni, ha avuto luogo la discussione e, su proposta del rappresentante del Governo, si è convenuto di rinviare il seguito dell'esame

degli organi di controllo e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili delle banche fallite, finalizzata ad adottare adeguate misure affinché, ove venga esercitata l'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2394*-bis* del codice civile nei confronti dei medesimi soggetti e ne risultino accertate le responsabilità, sia resa più agevole la facoltà di attivare le pene accessorie, con particolare riferimento all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero a stabilire l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 2) a realizzare in tempi rapidi una ricognizione del complesso delle norme sanzionatone, sia di rango penale che amministrativo, al fine di verificarne l'adeguatezza, tenendo conto del quadro normativo dell'Unione europea in materia, compresa, per quanto riguarda le banche beneficiarie di aiuti di Stato, la Banking Communication del 2013; 3) ad attuare nei tempi previsti le misure per la promozione e l'effettiva diffusione dell'educazione finanziaria - consentendo la piena operatività del comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, di cui al decreto-legge n. 237, convertito dalla legge n. 15 del 17 febbraio 2017 - allo scopo di aumentare la conoscenza da parte dei cittadini degli strumenti e dei servizi finanziari immessi sul mercato, nonché la loro capacità di valutazione dei profili di rischio associati alle diverse tipologie di prodotti offerti. tal fine ad assumere iniziative, con il coinvolgimento delle autorità nazionali di vigilanza, per garantire la corretta applicazione, da parte di tutti soggetti abilitati a prestare servizi di investimento, delle regole finalizzate ad impedire il collocamento degli strumenti finanziari più rischiosi presso clienti al dettaglio non in grado di comprenderne l'effettivo rischio, e al contempo a rafforzare le sanzioni per il mancato rispetto di tali regole; 4) a favorire, nell'ambito di quanto previsto dalle normative europee e dai criteri stabiliti dalla legislazione vigente, il posticipo del termine previsto per accedere al beneficio del ristoro; ristoro; 5) a istituire, in accordo con le istituzioni dell'Unione europea e nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, un veicolo speciale per assistere le banche nell'opera di pulizia dei bilanci, in grado di creare un mercato dei crediti deteriorati, il cui smobilizzo ordinato,

Signor Presidente, rispetto al testo che ho letto prima, d'intesa con tutti i Gruppi, sono state operate tre modifiche. La prima riguarda il primo capoverso dove, alla terza riga, è stata la tolta la parola «fallite» dopo la parola «banche».

Signor Presidente, le vicende bancarie sono state una specialità dei Governi succedutisi a partire dal 2014. Nel corso dell'ultimo biennio le vicende che riguardavano le banche hanno tenuto banco nel Paese e hanno avuto delle conseguenze oggettivamente difficili da gestire penalizzando la competitività dei nostri mercati e monopolizzando a più riprese l'attenzione del Governo. Un po' di storia non fa male. si è verificato a partire dalla pausa natalizia di due anni fa. Proprio allora, tra Natale e Capodanno, si è scoperto che quattro banche italiane, capeggiate da Banca Etruria, erano in *default* e che, al fine di salvarle e ricapitalizzarle, il Governo allora presieduto da Matteo Renzi, aveva ratificato in tempi *record* la direttiva europea sul *bail facendo particolare attenzione a salvare gli amministratori delle banche responsabili non solo della cattiva gestione, ma in alcuni casi anche di aver impartito direttive che avrebbero portato alla truffa di migliaia di piccoli risparmiatori, i quali sarebbero stati indotti, a loro insaputa, a investire in titoli obbligazionari altamente rischiosi. Tale solerzia da parte del Governo non fu allora utilizzata per rendere operativa la direttiva gemella che si occupava di proteggere i risparmi dei correntisti degli istituti in crisi, i quali si sarebbero altrimenti visti azzerare i conti. Qualche mese più tardi una sorte simile, con profili solo apparentemente meno grotteschi, è stata riservata alle banche venete, alla Banca Popolare di Vicenza e a Banca Carige, per le quali lo Stato italiano ha stanziato, tra garanzie e interventi, 20 miliardi di euro di denaro pubblico. Se le banche sono state salvate, i 200.000 piccoli azionisti, che erano stati persuasi a sottoscrivere azioni delle due banche come attività propedeutica alla concessione di un prestito, hanno pagato il prezzo più alto perdendo tutto ciò che avevano investito. Questi piccoli risparmiatori subiranno oltre al danno, la beffa. Infatti, se nel caso di Banca Etruria e delle altre tre si era deciso di mettere a disposizione, almeno sulla carta, rimborsi per i risparmiatori con investimenti fino a 100.000 euro, nel caso delle banche venete il trattamento non è stato nemmeno simbolicamente paragonabile. Non possiamo poi fare a meno di citare in questa sede un terzo caso, che si è insinuato tra i due: il caso di Monte dei paschi di Siena. Siena. Per Monte dei paschi di Siena abbiamo assistito a un *modus operandi* diverso nella forma e nella sostanza, sia dal primo che dal secondo caso. Nonostante l'istituto di Rocca Salimbeni fosse già ricorso al mercato per 8 miliardi negli ultimi due anni precedenti l'ultima iniezione di liquidità, si è di fatto verificato un nuovo fallimento, che è costato allo Stato - quindi ai contribuenti - ulteriori 20 miliardi. In questa occasione il Governo, dopo aver di fatto sostituito i vertici in carica con uomini di sua fiducia e aver affidato una consulenza a sei zeri a JP Morgan, ha trovato il modo di sfuggire - solo in questo caso e solo per Monte dei paschi - all'applicazione del *bail in*. Gli azionisti e gli obbligazionisti di Monte dei paschi, a differenza dei loro omologhi veneti, toscani, marchigiani e genovesi avrebbero potuto dormire sonni tranquilli. Per loro la via della salvezza era stata imboccata. Signor Presidente, signori del Governo, io credo che possiamo

bancario italiano è per ora salvo. Il prezzo che abbiamo pagato è stato un prezzo alto, in tutti i sensi.

di risultati di discutibile utilità. Ne faccio una brevissima sintesi. Uno, far pagare agli investitori, e in particolare agli obbligazionisti, le spese della mala gestione delle banche in questione. utilizzare tre pesi e tre misure ai danni dei risparmiatori: nel caso di Banca Etruria e delle altre tre banche sono stati garantiti rimborsi (per ora più simbolici che reali), nel caso delle banche venete nessuna garanzia è stata prevista e nel caso di Monte dei paschi si è garantita la protezione totale di tutti i conti e degli investimenti. proteggere i vertici delle banche in dissesto - in molti di questi casi palesemente responsabili della mala gestione dei conti - da eventuali responsabilità o da ipotetiche cause di risarcimento da parte dei risparmiatori. Quattro, permettere - a volte anche perché era l'unica strada praticabile - a vari soggetti privati di trarre benefici economici da questi *default*. Signor Presidente,

Credo anche - e mi avvio a concludere - che questo sia innanzitutto una vittoria di chi ha preso l'iniziativa. Devo dire che il nostro Gruppo, che ha presentato per primo è orgoglioso di averlo fatto. Ringrazio il senatore Augello per l'iniziativa assunta e ringrazio la senatrice Bonfrisco che con la sua competenza, soprattutto sulle banche venete, ha

può rappresentare una speranza, ma non una certezza e noi siamo abituati a preferire certezze rispetto a dati di fiducia, sopratutto nei confronti di un Governo che non la merita. Tuttavia, alla fine abbiamo deciso di ritirare la nostra mozione, che era più stringente e vincolante e conteneva maggiori punti a tutela dei risparmiatori e contro coloro che hanno creato questo dissesto e lo abbiamo fatto per un semplice motivo: perché vogliamo togliere ogni alibi al Governo rispetto ai contenuti di questo ordine del giorno. A fronte di questo gesto, di questa volontà di approvare un testo unitario, pretendiamo che in questo scorcio di legislatura il Governo onori

Sappiamo tutti che questa esigenza è nata quasi due anni fa con il famigerato e pessimo provvedimento salva banche, che ha eliminato il rapporto di fiducia tra risparmiatori, sistema bancario, politica e Governo;

Le responsabilità di tutte queste vicende, di questi dissesti e di queste truffe sono di duplice natura: da una parte, della politica, che non ha saputo agire per difendere il proprio sistema economico e di conseguenza bancario e, dall'altra, dei grandi dirigenti di questi istituti, che stanno godendo ancora dell'impunità, nell'inerzia del Governo che non approva leggi che invece li penalizzino. L'unica certezza è che in tutte queste vicende sono stati i cittadini a essere truffati, ad aver perso tutti i loro risparmi, con un atteggiamento incomprensibile del Governo che ha penalizzato maggiormente i risparmiatori di alcune banche rispetto a quelli di altre non ha saputo trovare soluzioni a tutela di azionisti e risparmiatori che hanno investito in obbligazioni le loro risorse. Ecco, questa è l'unica certezza: i risparmiatori sono stati penalizzati e i responsabili non hanno pagato. Noi vorremmo un modello diverso in cui il Governo tuteli i risparmiatori, si ponga questo obiettivo come primario e necessario, colpisca coloro che sono responsabili e cerchi di cambiare una politica che evidentemente non funziona. *(Applausi

ramo del Parlamento, rafforza il Governo in un compito non facile di confronto con l'Unione europea sul tema delle crisi bancarie. Infatti è innegabile, dovendo fare una fotografia di quello che è avvenuto negli ultimi anni, che vi siano stati, nelle diverse fasi, due pesi e due misure. certamente vi è stata una maxi-iniezione di denaro pubblico in molti Stati europei per il salvataggio delle banche mentre l'Italia, in quella fase, non scelse questo tipo d'intervento; successivamente, quando in occasione degli *stress test*, quindi della valutazione della capacità delle banche a resistere ad eventuali crisi sistemiche, sono stati fortemente sottovalutati i rischi connessi ai derivati tossici che si trovavano nella pancia di numerose banche, in particolare di quelle tedesche. Allo stesso modo, un occhio di riguardo è stato rivolto e continua a essere rivolto nei confronti delle casse di risparmio tedesche, che stanno conoscendo una crisi non molto dissimile da quella delle nostre banche minori. Credo, quindi, che esista un altro problema, che è già stato rimarcato. Nel nostro Paese abbiamo avuto tre strumenti di intervento: *burden sharing*, ricapitalizzazione e liquidazione coatta amministrativa.

ci voglia poco tempo per recuperare questo rapporto di fiducia, ma per farlo è necessario dare alcuni segnali chiari. Innanzitutto, con un pizzico di orgoglio posso dire che il primo punto dell'ordine del giorno G1 recepisce integralmente il senso e il significato dell'emendamento che presentammo alla Camera, che riporta all'idea che occorra tornare al principio fondamentale del «chi sbaglia paga» e, soprattutto,

e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili delle banche, finalizzata ad adottare adeguate misure affinché, ove venga esercitata l'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile nei confronti dei medesimi soggetti e ne risultino accertate le responsabilità, sia resa più agevole la facoltà di attivare le pene accessorie,

l'invito pressante al Governo è di trovare, nel più breve tempo possibile, il veicolo legislativo per poter passare da un impegno in un ordine del giorno a un atto normativo che possa essere più stringente. Il secondo aspetto che desidero evidenziare

del tutto solare che nella percezione dei risparmiatori occorra trovare un minimo comune denominatore che li tenga tutti assieme. Per queste ragioni, ringraziando ancora i colleghi e soprattutto il sottosegretario Baretta, il Gruppo Articolo 1-MDP

nel sottolineare l'esigenza di riformare e rafforzare il nostro sistema sanzionatorio e di controllo nei confronti degli istituti di credito, riteniamo che si debba proseguire nell'azione di tutela dei risparmiatori e dei detentori di obbligazioni, sia in riferimento

di determinare un percorso ordinato e sistemico di riduzione dei fattori di rischio e di sostegno alla stabilità finanziaria del nostro sistema bancario. Ciò che oggi riteniamo debba costituire oggetto di valutazioni responsabili da parte di tutti i Gruppi parlamentari è l'impegno, che noi intendiamo preservare, a far sì che la Commissione di inchiesta sul sistema bancario sia strumento di una riflessione sia in ordine ai fattori di criticità, come l'incidenza dei crediti deteriorati sui bilanci bancari, sia in relazione alle condotte illecite e fraudolente che hanno determinato il dissesto di diversi istituti di credito. Abbiamo tutti una evidente responsabilità politica nell'evitare che i lavori della Commissione di inchiesta, a maggior ragione in questa delicata fase di conclusione della legislatura, siano viziati da logiche di parte e di strumentale contrapposizione politica, in primo luogo, per essere ancor più espliciti, nei confronti della massima autorità di vigilanza rappresentata dalla Banca d'Italia. La indispensabile valutazione degli elementi di criticità e dei comportamenti illeciti deve avere, a nostro giudizio, una prospettiva fondamentale: indicare gli ulteriori interventi ritenuti necessari per porre il sistema in sicurezza, nel medio e lungo termine, e su queste basi operare affinché il confronto in sede europea affronti il tema di nuove regole per garantire il futuro dell'unione bancaria. Occorre, infine, rendere efficiente il nostro sistema bancario e ciò, prioritariamente, riguarda il sostegno a un

Il senatore Gasparri, con la chiarezza che gli si deve ogni volta che parla, ha presentato questa lettura, secondo me capovolta, di quanto avvenuto nel nostro Paese. La sua tesi è presto detta: la responsabilità del tracollo del prodotto interno loro, delle crisi economiche e delle banche è del Governo tecnico del presidente Monti, che ha arrecato danni maggiori - dice il senatore Gasparri - di quelli che avrebbe dovuto evitare. Ovviamente, il senatore Gasparri dimentica che nel gennaio 2011 lo *spread* era a 173 punti, che nel novembre dello stesso anno superava abbondantemente i 520 punti. Dimentica le liti permanenti di quell'anno all'interno della maggioranza e, soprattutto tra luglio e agosto, tra i ministri Tremonti e Brunetta. Gasparri dimentica la riscrittura di numerose manovre finanziarie che hanno dato il segno di un Governo Berlusconi piuttosto allo sbando, di una maggioranza divisa e in confusione; e dimentica anche che, nel contesto di un'economia reale che cominciava a battere in testa, proprio il mondo bancario è riuscito - grazie al cielo - a reggere a reggere la tempesta, avendo però in pancia titoli del debito di Stato italiano in misura superiore a quanto la prudenza consigliava agli stessi istituti di credito e si è evitato quel *default* finanziario che danni incalcolabili e tragici avrebbe prodotto sull'economia e sulla società italiana.

sulla valutazione del rischio di credito, ci sono stati comportamenti criminali nel rapporto con la clientela meno finanziariamente attrezzata e l'inadeguatezza di amministratori e del *management* nell'affrontare situazioni aziendali sull'orlo di crisi irreversibili. Certo, non è tutto così il sistema del credito in Italia e non è affatto tutto nero, ma è stato anche così; forse oggi meno di ieri, ma certamente in alcuni istituti di credito c'è stata una grave sottovalutazione dei problemi e soprattutto della gestione manageriale. A noi appare allora che la strada perseguita con quest'ordine del giorno unitario sia condivisibile, perché non è quella solo di coloro che vogliono l'aumento delle punizioni

rischio. Non pare sempre noto a tutti, infatti, che ad alti tassi d'interesse corrispondono maggiori rischi e che comunque, in ogni operazione finanziaria, anche quella apparentemente più sicura, c'è il rischio della perdita totale o parziale del capitale investito. Dopo l'Argentina, dopo la Grecia, dopo il caso Parmalat e di tante altre società, abbiamo ancora fasce della popolazione - di quella popolazione che risparmia - che ritengono l'investimento finanziario

responsabilità degli amministratori. Quell'emendamento nel decreto salva banche

il collasso di sette banche, altre in uno stato di grandissima difficoltà, oltre 50 miliardi di risparmi bruciati e almeno altri 50 miliardi di costo socializzato per favori fiscali,

di queste banche. Le regole europee pongono un limite ai *bonus* dei banchieri, ma il problema è che quando va bene, incassano, ma quando va male, non pagano. Questo è il problema che ci siamo trovati di fronte. Un consigliere Un consigliere su quattro nei consigli di amministrazione delle banche italiane quotate non è in regola, cioè non rispetta i nuovi vincoli BCE, vale a dire le norme introdotte dalla quarta direttiva europea

Si tratta di una pena opportuna nei confronti dei *manager* responsabili degli istituti di credito e di coloro che sono chiamati a rispondere in un'azione di responsabilità. D'altra parte, l'ipotesi

l'Esecutivo proprio in questa direzione, ovvero verso l'adozione tempestiva di una normativa sulla responsabilità degli amministratori delle banche fallite, con particolare riguardo alle responsabilità dei vertici aziendali. Insomma, facciamo un altro passo in quella direzione; si tratta comunque di passi piccoli,

in arrivo al Senato. Mi riferisco, ad esempio, a un impegno che prevedeva di valutare l'adozione di misure che garantiscano un equo trattamento di ristoro a tutti gli investitori coinvolti e penalizzati dai comportamenti illeciti nella gestione delle banche e che hanno causato la crisi del sistema bancario negli ultimi due anni. due anni. Ahimè, questo impegno è rimasto lettera morta. bancario - lo sottolineo: il sistema bancario - avrebbe dovuto sborsare 13 miliardi di euro per coprire il valore dei depositi da rimborsare tramite il Fondo interbancario di garanzia: ben 13 miliardi di euro. Il Governo ritenne allora di far risparmiare al sistema bancario quei 13 miliardi andando a chiedere ai cittadini italiani di sobbarcarsi l'onere e il rischio di pagare di tasca propria fino a 17 miliardi di euro solo per Veneto Banca e Popolare di Vicenza. la procedura di liquidazione ha tolto ai risparmiatori truffati la possibilità di chiedere un risarcimento in tribunale. Questo è bene ricordarlo, perché, pur in presenza di una sentenza che preveda un risarcimento, avendo il Governo regalato a Banca Intesa la parte sana delle due banche, non vi sarà capitale da aggredire per dare esecuzione alle stesse sentenze. Insomma, è stato dato un colpo di grazia agli oltre 200.000 piccoli azionisti che avevano acquistato, nell'arco degli anni, quote azionarie delle due banche.

In conclusione, stanti le premesse, esprimo voto favorevole del Movimento 5 Stelle all'ordine del giorno unitario. Tengo a puntualizzare che il punto 3) del dispositivo, quello relativo all'educazione finanziaria che viene auspicata in termini di aumento della conoscenza da parte dei cittadini degli strumenti finanziari, ci trova concordi in quanto l'intervento di per sé mira ad un aumento dell'educazione finanziaria nel nostro Paese, di cui c'è bisogno. Riteniamo, però, sia opportuno far presente che questa mancanza di educazione e di conoscenza degli strumenti finanziari non può e non deve essere attribuita ai cittadini, ai piccoli azionisti, ai risparmiatori che sono stati truffati, perché sono stati vittime non di un incauto acquisto, ma di truffe e raggiri, di falso in bilancio, di ostacolo alla vigilanza, di aggiotaggio, rispetto

il testo in esame come l'inizio di una politica diversa da parte del Governo, che fino ad ora abbiamo visto essere abbastanza timido su questa materia. Le dinamiche e gli esiti non compiuti relativi alla famosa Commissione d'inchiesta in materia testimoniano come ci sia stata non una volontà dilatoria, ma certamente un atteggiamento frenante da parte del Governo e della maggioranza ad entrare nel vivo di tali questioni.

delle norme vigenti non sia sufficiente, non tanto a punire i colpevoli di eventuali reati di

del voltarsi dall'altra parte, per evitare forse di intercettare comportamenti anomali da parte di persone vicine al vertice governativo. Ripeto, oggi speriamo inizi un atteggiamento diverso, dato che l'intero Parlamento accoglie e promuove l'ordine

inserisca un sollecito rivolto a se stesso, è significativo di quanto queste procedure siano lente e farraginose. Oggi come oggi l'unica educazione finanziaria che ha potuto

Molte migliaia di cittadini italiani si sono dovute educare sul campo al rischio che hanno subito nel sottoscrivere determinati prodotti finanziari e ciò ha prodotto anche un effetto di conoscenza. Credo che ormai tutti gli italiani che si recano presso le banche o gli intermediari finanziari a sottoscrivere nuovi prodotti siano molto più accorti o, quantomeno, abbiano un'ansia di approfondimento dei possibili rischi del prodotto che vanno a sottoscrivere, che non rappresenta già una salvaguardia, ma che certamente consente loro un atteggiamento di maggiore prudenza.

ancora una volta in Europa, per chiedere una deroga, ove necessario, alle attuali normative. Quindi, porre l'accento sulle procedure è importante, perché autorizza il Governo ad attivare questo tipo di

raggruppano diverse fattispecie di crediti (da quelli in sofferenza ai dubbi esiti agli incagli), hanno certamente un'incidenza forte sui bilanci delle banche e sul sistema finanziario complessivo, hanno anche una refluenza estremamente importante sull'economia reale, perché in questo momento in cui ancora permangono gli effetti della crisi - per quanto

un'unica categoria da gettare nel cestino o da affidare ai cosiddetti riscossori coattivi fuori dal sistema bancario, ma vanno gestiti con accortezza nell'ambito dello stesso sistema bancario, perché le banche non possono scaricare

proposto dal Governo e dalle altre forze politiche. signor Sottosegretario, si può dire che per una volta ci troviamo ad affrontare la complessa questione bancaria senza il vizio di uno strabismo elettorale che molte volte, purtroppo, ha connotato un confronto su questo tema importante e delicato. Senza questa forma di strabismo, si è potuto porre invece l'accento sul ruolo del cittadino risparmiatore. Nel caso di queste mozioni, tutto prende le mosse dal decreto-legge n. 99 del 2017, che rappresenta un ulteriore e decisivo passo per la stabilizzazione del sistema bancario, dopo l'intervento fatto sulle quattro banche poste in risoluzione e dopo la ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi di Siena a fronte del risultato negativo di uno *stress test* condotto in condizioni avverse.

per interventi fatti sulle singole banche. Noi siamo riusciti ad evitare di ricorrere a questo strumento, ma una riflessione sull'equilibrio che ci deve essere fra questi due meccanismi è assolutamente necessaria. la 6a Commissione, infatti, è in corso un'ampia ed approfondita analisi delle proposte volte a modificare il *bail in* stesso

essere presenti ai tavoli, e quindi affrontare questo tema in fase ascendente, dando un ruolo al Parlamento italiano nel processo legislativo europeo. Penso che ciò rappresenti

per fare una riflessione seria e compiuta, che coinvolga tutto il Senato e non solo la Commissione, su un tema importante e delicato. Oggi però, fondamentalmente, si è raggiunto un buon risultato grazie al combinato disposto e all'interazione tra il lavoro parlamentare e la disponibilità del Governo, che qui ringrazio. Sicuramente un voto unanime, come quello che si sta profilando, ha il vantaggio, importante e significativo, di rafforzare l'azione del Governo nell'interlocuzione con l'Unione europea. Prima ho citato i tre strumenti utilizzati

che acquisire in maniera forte una maggiore solidità sia un salto di qualità anche nella nostra capacità di stare intorno a quei tavoli. Allo stesso modo, come emerso anche nelle indagini conoscitive, importante battersi perché ci sia una diversa valutazione del rischio di mercato rispetto al rischio di credito anche a favore delle nostre banche. Ad ogni modo, con l'ordine del giorno in esame abbiamo ottenuto un doppio risultato, rafforzando il Governo nell'interlocuzione con l'Unione europea, ma anche - penso dando un contributo significativo per rimettere in moto un processo di fiducia dei cittadini nei confronti del mondo bancario, essenziale a fronte della rivoluzione copernicana rappresentata dall'introduzione del *bail